la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 14 novembre 2007. L'ordine del giorno di oggi è stato integrato, a partire dalle ore 12, con la discussione delle mozioni sull'attribuzione dei seggi italiani al Parlamento europeo. Dopo le illustrazioni, Dopo le illustrazioni, per cinque minuti, potranno intervenire i Gruppi per cinque minuti ciascuno (dieci minuti al Gruppo Misto). Per quanto riguarda gli altri argomenti all'ordine del giorno di oggi e domani, la Conferenza ha proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi per il decreto-legge sull'avvio dell'anno scolastico e per il seguito della discussione dei disegni di legge di assestamento e rendiconto. Quest'ultima riprenderà oggi pomeriggio a conclusione del decreto-legge o, in ogni caso, in apertura della seduta antimeridiana di domani. Al fine di consentire il completamento dell'esame dei provvedimenti in questione entro la settimana corrente, la seduta antimeridiana di domani potrà protrarsi oltre il consueto orario e l'esame di merito potrà proseguire anche nel pomeriggio, ove non concluso. Il Parlamento in seduta comune è convocato oggi alle ore 11 per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi i deputati, cosicché la chiama dei senatori abbia inizio attorno alle ore 13. Nel corso della prossima settimana sarà discusso il decreto-legge in materia economico-finanziaria, per il quale pure si è proceduto alla ripartizione dei tempi per complessive venti ore, al fine di assicurare il voto finale entro la giornata di giovedì 25 ottobre. La Conferenza dei Capigruppo ha poi definito gli ulteriori tempi della sessione di bilancio. La 5a Commissione permanente dovrà concludere l'esame dei documenti finanziari entro mercoledì 31 ottobre. L'Assemblea non terrà seduta nel corso di tale settimana. L'esame in Aula avrà inizio nella seduta pomeridiana di lunedì 5 novembre e proseguirà per tutta la settimana fino a venerdì 9, per riprendere la settimana successiva dal pomeriggio di lunedì 12 e concludersi entro la giornata di mercoledì 14 novembre. I tempi sono stati ripartiti per complessive cinquantasei ore. Infine, la Conferenza dei Capigruppo ha concesso all'unanimità la deroga per l'esame, durante la sessione di bilancio, del disegno di legge n. 1628 concernente la ratifica dell'accordo sui brevetti europei. Il calendario potrà essere pertanto integrato con tale provvedimento, non appena concluso dalla Commissione competente. Nel periodo compreso dal calendario saranno altresì svolte interrogazioni urgenti sul caso De Magistris.

Un dramma sociale che potrà ancor più aggravarsi e acutizzarsi se cadrà nel silenzio, se verrà rimosso e censurato, se le forze democratiche e le istituzioni della Repubblica lo ignoreranno. Signor Presidente, da alcuni giorni a Cosenza 35 famiglie stanno occupando uno stabile al centro della città, in uno dei quartieri più poveri e popolari di Cosenza. Diverse famiglie, colleghe senatrici, colleghi senatori, vivono in case già dichiarate da tempo inagibili. Molte, con i loro figli, vivono in vere e proprie topaie; altre vivono in case angustissime, angustissime, con i bambini costretti a vivere, giocare, dormire nelle cucine, nei corridoi, nelle camere da letto dei genitori. Tutte queste 35 famiglie, assieme a tante altre di Cosenza, attendono invano da circa un ventennio non solo una casa, ma una qualsiasi risposta da parte di tutte le varie amministrazioni politiche che si sono succedute a Cosenza. E persino le graduatorie per gli alloggi - il minimo democratico - sono introvabili a Cosenza. Ieri, signor Presidente, sono stato nello stabile occupato: occupato: asserragliate, nel buio e nel freddo, vi sono oltre 100 persone tra cui tante donne, giovani e anziani e 30 piccoli bambini, dai due agli otto anni. Non voglio fare - non serve - nessun esercizio retorico. Ma sui volti di tutto loro è impressa una grande sofferenza sociale,

specialmente agli esponenti del Partito Democratico - perché sarebbe vergognoso che il nascituro partito si presentasse così in Calabria - un'assunzione di responsabilità. Lo sgombero violento di questa notte va evitato e va aperta

Nella seduta precedente, su questo argomento avevo rivolto al Governo una precisa richiesta, di cui lei, signor Presidente, si era fatto carico, nei confronti sia del Presidente del Consiglio che del Ministro dell'economia. La richiesta era quella di far conoscere all'Aula come mai, avendo il Governo più volte indicato un maggior gettito per il 2007, stimato in circa 25 miliardi di euro,

che perseguitano i cittadini. Siamo arrivati al punto che in città come Roma e Napoli, per un credito di 1.800 euro risalente ad una presunta contravvenzione di quindici anni fa, c'è il pignoramento di beni mobili e immobili.

il provvedimento al nostro esame reca «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari» e giunge a noi dalla Camera dei deputati dopo un proficuo lavoro emendativo, sia nelle Commissioni (VII e XI), sia in Aula. Si tratta di un provvedimento di urgenza volto a rendere più efficace l'attività della scuola dando certezza normativa e maggiore funzionalità ad alcuni punti specifici, ma significativi, della sua organizzazione e dei suoi procedimenti. Tali interventi rispondono, a nostro parere, ad esigenze sentite delle famiglie, della società e della scuola. Un articolo - l'articolo 3 - riguarda l'assunzione di ricercatori e risponde anch'esso a ragioni di necessità e di urgenza. All'articolo 1, comma 1, si reintroduce nella scuola primaria l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Nella storia della scuola italiana degli ultimi trent'anni l'esperienza del tempo pieno rappresenta un punto chiave nella realtà educativa e sociale del Paese e uno degli aspetti più innovativi dell'organizzazione didattica.

alla necessità dell'integrazione dei disabili e dei minori in difficoltà, ai comportamenti problematici dei ragazzi e dei preadolescenti, di fronte alla sfida storica dell'immigrazione dei minori stranieri nel sistema di istruzione nazionale, costruisce una grande scelta politica. È ben vero che questo intervento è qui previsto senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma la legislatura è agli inizi e noi confidiamo che maggiori risorse finanziarie e organizzative possano in altra sede essere previste. Il provvedimento prevede la definizione di un piano triennale di intervento da parte del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza unificata, al fine di incentivare e sostenere su tutto il territorio nazionale, e in particolare nel Mezzogiorno, l'esperienza del tempo pieno e del tempo prolungato. una scelta positiva adottata nei confronti dei ragazzi e delle famiglie, sollecitata anche da proposte di legge di origine parlamentare, che, siamo certi, concorrerà a migliorare la qualità della scuola italiana, il suo profilo culturale ed educativo, la coesione sociale del Paese. 1 introduce norme più rigorose per l'individuazione della sede d'esame dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria superiore. La scelta sarà operata non più dai candidati privatisti, ma dal dirigente scolastico regionale sulla base delle preferenze espresse dai candidati, assegnando gli stessi ad istituti statali o paritari del Comune di residenza, della Provincia, della Regione. Il comma 3 fissa i limiti di spesa per la corresponsione dei compensi per gli esami di Stato conclusivi della istruzione secondaria superiore in 183 milioni di euro dal 2007, elevando di 45 milioni l'importo già previsto dalla legge finanziaria del 2007. Al comma 4 viene ripristinato il giudizio di idoneità o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo della scuola media di primo grado da parte del consiglio di classe e viene prevista una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento. Il comma 5 riduce da otto a tre i componenti del comitato di indirizzo dell'INVALSI, esperti di qualificata competenza sulla valutazione nazionale e internazionale, di cui uno proveniente dal mondo della scuola. Nello stesso comma si affida al Ministro della pubblica istruzione l'emanazione della direttiva annuale con l'indicazione degli obiettivi della valutazione esterna prevista per gli studenti di seconda e quinta classe per la scuola primaria, di prima e terza media, di seconda e quinta classe superiore. Il comma 7 autorizza la spesa necessaria di 9.783.656 euro per il funzionamento delle "sezioni primavera", da ventiquattro a trentasei mesi di età, che ampliano l'offerta educativa nei primi anni dell'infanzia del nostro Paese, anche con iniziative sperimentali sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica e flessibilità. Nello stesso comma si riconoscono come titoli abilitanti per gli insegnanti nelle scuole paritarie dell'infanzia i diplomi conseguiti presso le scuole o gli istituti magistrali. L'articolo 2 prevede norme urgenti in materia di personale scolastico. Interviene in materia di sanzioni disciplinari, di sospensioni cautelari, di trasferimenti per incompatibilità ambientale, prevedendo procedure semplificate e più veloci e la responsabilizzazione del dirigente scolastico. Si tratta di una materia delicata poiché riguarda i comportamenti del personale della scuola e la qualità professionale dei docenti che sono la prima garanzia per la stessa qualità della scuola. Il risalto mediatico dato alla cronaca spesso amplifica i fatti rendendo ancora più necessaria la tutela delle persone coinvolte, a cominciare dai più indifesi. Sono in gioco la tutela dei minori e del loro diritto all'istruzione, l'interesse delle famiglie ad un servizio scolastico di qualità e la loro fiducia nella scuola, la serietà dei comportamenti del personale, la tutela del diritto individuale alla difesa. Il parere sul punto della 1a Commissione è importante. Dopo avere espresso, per quanto di competenza, parere non ostativo, la Commissione affari costituzionali del Senato ha invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di garantire nelle procedure di irrogazione delle sanzioni, disciplinate dall'articolo 2, il necessario rispetto del principio del contraddittorio, richiamando altresì la inviolabile libertà di insegnamento garantita dall'articolo 33 della Costituzione. Se è doveroso intervenire per assicurare alla scuola serenità ed efficacia, è altrettanto necessario farlo non ristringendo l'orizzonte della ricerca di livelli più elevati della convivenza nel segno del rigore morale, della trasparenza, del rispetto dei valori costituzionali. Lo stesso concetto di incompatibilità ambientale è oggi soggetto ad una più approfondita interpretazione se si considera il ruolo della scuola anche rispetto ai condizionamenti del contesto. Il comma 3 dello stesso articolo consente ai dirigenti scolastici di provvedere direttamente al conferimento delle supplenze dei collaboratori scolastici, snellendo le procedure. Il comma 4 modifica opportunamente i termini per la comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro da parte delle istituzioni scolastiche, ovviando alle difficoltà riscontrate al riguardo, mentre il comma 5 dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, l'imputazione a carico dei capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione delle spese relative alle supplenze di maternità, integrando detti capitoli di 66 milioni di euro per il 2007 e di 198 milioni a decorrere dal 2008. Questo intervento libera risorse importanti per la scuola. L'articolo 3, infine, reca - come si è detto - disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori consentendo l'utilizzazione delle somme previste per l'anno 2007 e assegnandole al Fondo per il finanziamento ordinario delle università e al Fondo di finanziamento per gli enti di ricerca. L'assunzione dei ricercatori prevede concorsi regolati dalla disciplina vigente, nonché, per l'attività scientifica e didattica, la valutazione triennale; un primo passo per il necessario rapporto tra la qualità dell'attività e l'assegnazione delle risorse. Signor Presidente, l'urgenza del provvedimento all'esame e la ragionevolezza dei suoi interventi consigliano - a nostro parere - una sua rapida approvazione da parte dell'Aula del Senato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è qualcosa di drammaticamente velleitario in un Ministro della pubblica istruzione che afferma di voler tracciare il futuro ma con il capo volto all'indietro e lo sguardo fisso a scelte ideologiche del passato; che annuncia un ritorno alla serietà e al rigore, non preoccupandosi però di proporre strumenti atti ad affermare concretamente tali principi; e che punta a cambiare la scuola non sulla base di un progetto definito, bensì di interventi occasionali dettati esclusivamente dall'urgenza, i quali obbligano poi il Parlamento ad operare con difficoltà e in condizioni di emergenza. Emblematico dello spirito velleitario "alla Fioroni" è in questo senso il decreto che il Senato è oggi chiamato a convertire in legge, un decreto-legge che peraltro arriva qui, in Aula, ad anno scolastico abbondantemente iniziato. Tale provvedimento, all'articolo 1, reintroduce il tempo pieno ma lo fa mantenendo inalterati sia gli organici che gli oneri di spesa, con il rischio di determinare paradossalmente una riduzione delle ore di insegnamento più che un loro aumento. E lo fa senza una preventiva revisione dei contenuti didattici e dell'organizzazione docente, con il rischio di imporre nostalgicamente un modello in realtà già superato. Il che può forse soddisfare coloro che, alla funzione formativa e responsabilizzante della scuola, preferiscono ancora quella meramente assistenziale, ma non certo le famiglie che, preoccupate per l'avvenire dei loro figli, guardano allo stato reale delle competenze e degli apprendimenti di base. Non solo. Il provvedimento tende anche a far passare per una specie di ripristino degli esami di riparazione quella che in una realtà è una diversa modalità del recupero dei debiti scolastici, tanto più che, per realizzare la suddetta variazione, si sarebbe resa necessaria una apposita modifica legislativa. Sempre all'articolo 1 del provvedimento in discussione si fa inoltre riferimento alle competenze delle Regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa. Ma vi sono Regioni, come la Toscana, che non danno corso alla formazione professionale, facendo ricadere tutto sul bilancio degli uffici scolastici regionali e privando così gli studenti di una adeguata offerta formativa professionalizzante. Per non parlare del fatto che un aspetto fondamentale riguardante la formazione professionale, legato all'innalzamento dell'obbligo scolastico dopo le medie, viene interpretato dalle Regioni - peraltro contro il dettato della legge - come una occasione per ridurre o addirittura sospendere i finanziamenti alla formazione professionale scaricando tutto sulle scuole. Da una indagine sui centri di formazione professionale (pubblicata in questi giorni) risulta - ad esempio - che la mia Toscana sia tra quelle Regioni che hanno inteso il biennio come esclusivamente scolastico, ignorando il passaggio che stabiliva il mantenimento dei percorsi professionali. All'articolo 2 si prevedono procedure sanzionatorie nei confronti di insegnanti inadeguati, i cui comportamenti creano problemi di incompatibilità ambientale. È una risposta all'emergenza educativa che sta caratterizzando anche quest'anno scolastico, ed è un modo per scardinare un sistema di tipo corporativo che, in nome del principio dell'autotutela, ha finito troppo spesso con l'accordare eccessive garanzie a docenti immeritevoli. Ma allora, trattandosi di sanzioni disciplinari che pongono in ogni caso il problema del tipo di garanzie, non sarebbe stato più opportuno rivedere lo stato giuridico degli insegnanti? E non sarebbe semmai il caso di introdurre - seguendo un progetto già avviato dall'ex ministro Moratti - un codice deontologico dei docenti? Non si può non apprezzare il "giro di vite" sui docenti che, per incompatibilità ambientale, costituiscono un ostacolo per il buon apprendimento. Ma non si può non osservare che tale provvedimento rappresenta uno strumento destinato ad intervenire solo in casi eccezionali, rari. Resta perciò la domanda: a quando un sistema veramente competitivo e autonomo, capace di dare ai dirigenti scolastici, come avviene nel resto d'Europa, la possibilità di assumere e licenziare in base ai risultati? A quando un sistema scolastico capace di prevedere retribuzioni differenziate e calibrate in base alla professionalità dei docenti? A quando, insomma, un sistema scolastico capace di valutare non solo le patologie, ma anche le eccellenze dei docenti? Solo un sistema fondato sulla meritocrazia e sulla valutazione legata ai risultati - e che veda le famiglie depositarie del loro diritto di scelta - potrà infatti

va rilevato, a proposito del comma l-*bis*, che è gravissimo attribuire all'ANVUR (il cui *iter* istitutivo è assai lungo) il compito di valutare i singoli docenti-ricercatori, anziché le sedi e i sistemi universitari. Ciò contrasta infatti con l'articolo 33 della Costituzione, che garantisce quell'autonomia universitaria comprensiva anche del reclutamento, della carriera e della verifica dei docenti. Vi è inoltre il rischio oggettivo che una verifica centralistica sulla qualità dei singoli ricercatori finisca per rivolgersi alla loro appartenenza politica. Infine, è ridicolo attribuire una verifica del genere ad un'agenzia che deve essere ancora definita e realizzata; affidare un'ingiusta valutazione ad un'agenzia inesistente è francamente il colmo del velleitarismo! Concludo, dati i tempi assegnatimi, suggerendo al ministro Fioroni un fioretto: lasci perdere il fanciullesco «gioco del cacciavite», col quale - come in un meccano - si diletta a scomporre e ricomporre la riforma Moratti e pensi semplicemente a svolgere il suo lavoro di Ministro della pubblica istruzione, dando magari certezze agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti, e riportando per davvero, con i fatti e non solo a parole, serietà e rigore nell'ordinamento scolastico italiano che, complice una generale caduta di valori della società, appare oggi profondamente degradato proprio nella sua duplice funzione primaria di formazione e di socializzazione.

Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, non mi soffermerò sugli elementi molto positivi contenuti in questo decreto, come il tempo Basti ricordare il valore di questo intervento dal punto di vista sociale ed educativo: uno strumento capace di costruire una scuola migliore e di venire incontro alla domanda di autonomia delle donne che lavorano. Anche altri provvedimenti sono positivi, come l'esame di terza media, la riorganizzazione dell'INVALSI, le risorse per gli esami di Stato e la definizione migliore della norma contro i cosiddetti Altre misure, come la valutazione dei ricercatori e le sanzioni nei confronti degli insegnanti, si sarebbero invece dovute collocare in una diversa sede normativa, consentendo così un dibattito più approfondito e soluzioni più avanzate. A proposito di questo primo provvedimento (cioè quello relativo ai ricercatori), mi auguro che la materia della valutazione sia rapidamente e complessivamente rivista, senza improprie accelerazioni. A proposito delle sanzioni, credo necessario un intervento complessivo di riordino degli organi collegiali, luogo dell'equilibrio tra i soggetti che vivono e lavorano nella scuola; riordino nel corso del quale dare compiuta forma alle questioni disciplinari. Per quanto riguarda l'università, l'ipotesi che la qualità dell'attività del singolo ricercatore sia sottoposta dopo tre anni a valutazione e che questa valutazione sia addirittura svolta da un soggetto ancora costituendo, non mi pare la proposta adeguata per costruire quell'università del merito che tutti noi vogliamo. Per quanto attiene alla scuola, la questione delle sanzioni per il personale docente, posta in un decreto per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, indebolisce secondo me quella fiducia che dobbiamo dare agli insegnanti proprio quando la società affida loro grandi responsabilità. Valorizzare la funzione e la dignità sociale degli insegnanti significa investire sul futuro delle giovani generazioni e sul destino del Paese. Possiamo immaginare che questi interventi siano stati introdotti sull'onda della cronaca, ma spesso la cronaca è cattiva consigliera, soprattutto quando non risponde al principio di realtà. Noi legislatori, invece, dobbiamo avere la consapevolezza degli effetti di lungo periodo delle scelte che introduciamo nell'ordinamento. Gli insegnanti e i giudici sono le uniche figure della pubblica amministrazione che, rispetto alle sanzioni sulla propria attività professionale, vengono giudicate anche da soggetti loro pari. Questo avviene in causa di un preciso dettato costituzionale: i giudici in ragione della necessaria terzietà del potere giudiziario e gli insegnanti per assicurare il rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita. Le motivazioni storiche di questa scelta dei padri costituenti sono note: troppo fresca era la memoria delle leggi razziali e dell'obbligo di iscrizione al Partito fascista nelle scuole e nelle università. In particolare, sull'incompatibilità ambientale sarebbe stato necessario un altro approccio. Si deve tener conto del delicato equilibrio che si instaura tra docente e discente e di come il contesto, anche familiare, non sempre operi per valorizzare il ruolo dell'insegnante e dell'educatore. Allora noi abbiamo il dovere di assicurare alla scuola ed agli insegnanti autonomia da ogni indebita pressione che il contesto possa esercitare, riconoscendo loro il ruolo fondamentale, tanto nella crescita culturale dei ragazzi quanto nella funzione educativa. Vogliamo una scuola radicata nel territorio, ma non subalterna ad esso. Forse sarebbe stato incompatibile anche quel prete che ha lasciato scritto: «Non ho seminato che contrasti, discussioni, contrapposti schieramenti di pensiero. Ho affrontato le anime e le situazioni con la durezza che si addice al maestro». Quel prete era don Milani.

non ha nulla di urgente come dal titolo, ma non fa altro che recuperare alcune misure previste dal decreto Bersani, che ha subito una battuta d'arresto per mancanza di adeguate coperture economiche. Quindi di urgente non c'è nulla. Altre iniziative potrebbero essere ritenute urgenti, ma le dirò alla fine. Nessuno urgenza dunque; semmai l'unica urgenza di cui possiamo parlare con fondatezza è l'inadeguatezza di questa compagine a governare questo sfortunato Paese. All'articolo 1 si tenta di ripristinare il vecchio modello del tempo pieno, con molte ambiguità e limiti. Viene ristabilita l'esistenza del modello di un tempo pieno per finta, limitandolo di fatto alle sezioni già esistenti e, forse, neppure a quelle! Infatti, la proposta non legittima la formula vera e completa ed educativa del tempo pieno, in cui crediamo. Il problema essenziale che limita l'applicazione del tempo pieno sono le compresenze. E queste, in virtù della diminuzione dell'organico delle nuove scuole, vengono bruciate per mantenere il totale di ore in classe e per far fronte alle diverse emergenze non coperte da risorse ordinarie. Non a caso la norma prevede la realizzazione del modello a tempo pieno pieno «nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto». Il Governo continuerà a dire nelle vetrine mediatiche di aver ripristinato il tempo pieno, ma con la finanziaria 2007 e quella in preparazione si continuerà ad erodere personale docente e ad evitare incompatibilità di bilancio. Con la clausola di salvaguardia, infatti, è stata determinata la riduzione del 60 per cento dei fondi di funzionamento delle scuole. Le scuole che hanno istituito il tempo pieno dovranno scegliere se rinunciare alla compresenze o utilizzare illegittimamente ore del sostegno o dell'attività alternativa alla religione cattolica o, infine, chiedere ai genitori di togliere un pomeriggio ed affidarlo alle cooperative sociali. Si tratta di opzioni già operanti che questa norma sottintende e sostiene. Quanto al rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola e della legge di bilancio, non si capisce come mai non si faccia riferimento all'aggregato alla finanziaria pubblica, dal momento che le disposizioni in esame investono anche la competenza degli enti locali. L'impressione è che il Governo voglia mettere in atto una politica degli organici non rigidamente calcolata sul rapporto frontale alunni-docenti, coinvolgendo Regioni e Comuni nell'organizzazione delle classi funzionanti a tempo pieno, nonché nello stanziamento di risorse finanziarie integrative, in quanto lo Stato potrebbe chiedere agli Enti locali il personale educativo per garantire i servizi connessi all'attuazione dell'orario settimanale di 40 ore per gli studenti abili e quelli diversamente abili, nonché per attività di integrazione di minori immigrati. Il comma 3 fissa, infine, in 178,2 milioni di euro per l'anno 2007 la spesa per gli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore. Mancano all'appello 45 milioni di euro. di euro. Lo avevamo detto, ci verrebbe facile dire! Il tutto per un esame che non conclude un ciclo programmato, ma in via di definizione ed il tutto per un esame che non ha nulla di nuovo, di innovativo rispetto all'esame precedente. Quindi, uno spreco in più. Alla fine questo è! Viene specificato nella relazione tecnica che sono a carico dello Stato anche i compensi per commissari esterni e per i presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, escludendo da tale compenso i commissari interni, che saranno quindi a carico delle scuole paritarie. L'aumento dei costi, infine, non viene coperto con risorse aggiuntive, bensì con la riduzione degli stanziamenti previsti dalla finanziaria 2007 per ambiti di intervento che qualificano l'offerta formativa, quali: l'obbligo scolastico, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la gratuità dei libri di testo, l'IFTS (il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore) e le innovazioni tecnologiche. Per quanto concerne l'istituzione delle cosiddette sezioni primavera, il Governo estende al Paese il modello dell'Emilia-Romagna, costoso per le famiglie meno abbienti. Il Governo di centro-destra aveva cercato di risolvere il diritto all'infanzia di tutti i bambini anticipando l'ingresso nella scuola a due anni e mezzo dei bambini che ne avevano le capacità riconosciute. Ma la costituzione di sezioni cosiddette primavera sembra assolvere all'unico scopo di nascondere il rifiuto politico dell'anticipo contenuto nella cosiddetta In realtà, con questa iniziativa, si determinano le seguenti situazioni: si amplia l'anticipo di un anno intero di età; le classi primavera verranno costituite con bambini di due anni; si destinano maestre statali (non si sa in quale modo - se, ad esempio, con il volontariato - e con quale procedura e tipo di pagamento) a queste sezioni, quando si contestava che le stesse potessero occuparsi di bambini di due anni e mezzo; si invade una competenza specifica degli enti territoriali (delle Regioni (delle Regioni e dei Comuni, in particolare) relativa agli asili nido, e, così si contraddice il giusto orgoglio del Governo di attuare un piano per la realizzazione di asili nido su tutto il territorio nazionale. In sostanza, si tratta di una statalizzazione di un pezzo degli asili nido, al quale verranno applicati gli insegnamenti, le regole, le metodologie, il calendario, le cattedre e gli orari della scuola dell'infanzia, che invece, con la legge n. 53 del 2003, venivano riservati esclusivamente ai bambini che si sentivano pronti a questo modello di istituzionalizzazione. Il tempo mi impedisce di approfondire le questioni riguardanti le sanzioni disciplinari agli insegnanti e l'assunzione dei nuovi ricercatori, su cui interverrò in fase di illustrazione degli emendamenti e di dichiarazione di voto.

In modo particolare, manca una regolarizzazione per le scuole di quelle tasse comunali e locali che per ora non vengono pagate, o sono pagate in misura ridotta o creano dei contenziosi. Non è poi stata attivata un'esenzione del pagamento IVA sul materiale didattico e sulla strumentazione didattica per le scuole, anche, per esempio, per l'acquisto di strumenti musicali e la formazione artistica dei ragazzi. inoltre, istituito un fondo *ad* *hoc* per ripianare i debiti pregressi delle scuole e le spese sostenute per garantire il diritto allo studio. Non viene attivata, infine, la modifica dello statuto dell'insegnante per la valorizzazione della funzione docente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, non voglio approfittare di questa discussione sul decreto-legge, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinario avvio dell'anno scolastico, per parlare di tutte le problematiche dell'universo scuola. La tentazione, in verità, è grande, perché non ci vengono offerte molte occasioni per parlare di scuola, soprattutto non ci vengono offerte occasioni per trovare o comunque proporre soluzioni secondo la nostra esperienza e il nostro orientamento politico. Non voglio rincorrere il Governo e il Ministro della pubblica istruzione sul loro terreno, quello delle cose che fanno, degli *scoop*, delle molte che potrebbero fare e che non realizzano e di quelle grazie alle quali si disfà quanto precedentemente costruito. Quest'ultima categoria risulta essere al momento la più consistente e ricca di interventi. Proprio per queste ragioni, però, prendo semplicemente atto, e con favore, della disponibilità del ministro Fioroni ad avviare una discussione generale sullo stato della scuola nella Commissione competente. Mi auguro che questa condivisione a tutto campo serva a produrre una seria e pacata riflessione e porti a qualche conclusione concreta. Vedremo dal tono del dibattito quale sarà la reale intenzione del Governo a non lasciare il Parlamento fuori da ogni scelta, come ha fatto finora. Vedremo se riusciremo, con la politica dei partiti e del Parlamento, ad uscire da una visione della scuola che sembra irrimediabilmente consegnata alle *lobby*, sindacati e burocrazia in testa. Vedremo se il ministro Fioroni vorrà essere un po' più il Ministro della Repubblica e quindi di tutti i cittadini, studenti e famiglie in modo particolare, quelle famiglie e quegli studenti che tutto il Parlamento rappresenta, o sarà di più il Ministro dei dirigenti, dei direttori generali, delle federazioni sindacali. Va ristabilito un primato in questo servizio, va rovesciata una visione. Se vi orienterete in questa nuova direzione, troverete nell'UDC un soggetto dialogante; se invece rimarrete nella vecchia ottica, senatrice Soliani, l'UDC sarà un durissimo oppositore. Non vogliamo avere pregiudizi, anche se quello che abbiamo visto finora, a cominciare dalla riforma dagli esami di maturità, non ci è piaciuto per nulla. Comunque, ci teniamo a fare un'opposizione seria. Un giornale molto vicino al centro-destra, ma anche molto libero nella sua linea editoriale, ha recentemente attaccato l'opposizione e il suo *leader* perché, dice il giornale, sarebbero solo capaci di denunciare, senza avanzare serie proposte alternative. Sono pienamente d'accordo con questo libero quotidiano, anche se l'UDC respinge la critica, poiché non è il nostro caso. In questo, come in altri settori, ci siamo sempre assunti la piena responsabilità, appunto facendo proposte. Per questa circostanza, per questo decreto, diciamo responsabilmente che l'avvio dell'anno scolastico non può essere ordinatamente disposto con un decreto-legge, che deve essere approvato senza il tempo di un'adeguata discussione e senza l'opportunità di possibili e necessarie variazioni. Non si può governare la scuola con i decreti-legge blindati. Chiediamo pertanto al Ministro, ma anche alla maggioranza che lo sostiene, che, una volta approvato questo decreto, ci si possa tornare sopra con libertà e ampia possibilità di giudizio. Le nostre preoccupazioni, infatti, partono da situazioni molto concrete: l'autorevolezza dei docenti, tanto per cominciare, che è fortemente minata e in alcuni casi gravemente pregiudicata, l'incertezza delle modalità di reclutamento e assunzione degli insegnanti, la scarsa reale autonomia didattica, limitata da infinite direttive, una cultura del disimpegno e della contestazione. Sono tutti frutti di una cultura di sinistra figlia del Sessantotto, che hanno prodotto gli attuali risultati. Altro che scuola come missione, altro che la figura dell'insegnante povero ma felice e onorato di svolgere un ruolo così importante per i suoi ragazzi! Lo snodo è tutto lì, cari senatori della maggioranza, dovete dimostrare di rinunciare in modo definitivo a quella cultura che ha sfasciato non solo non solo la scuola, ma anche altri settori della pubblica amministrazione. Dovete fare una seria autocritica, dovete arretrare, facendo arretrare burocrazia e sindacato nelle scelte della scuola, cominciando a guardare veramente gli interessi dei ragazzi, ad esempio con il rendere la famiglia soggetto principe nei processi organizzativi e decisionali. Rovesciare una visione significa appunto passare dalla visione dello studente operaio, figlia del Sessantotto, che produce cultura per la grande azienda di Stato, a quella dello studente figlio, che si forma per la vita secondo una morale, che acquisisce la necessaria professionalità per essere autonomo e capace di fare e di dare in modo creativo nel mondo del lavoro. Oggi, invece, la famiglia è l'appendice ultima alla quale viene solo concesso l'onere di pagare le scelte fatte da altri. in questo pagare non mi riferisco solo a situazioni di tipo morale o educativo, ma anche a situazioni molto concrete di rilevanza economica. Infatti, la presunta gratuità della scuola dell'obbligo fino ai 16 anni si è in realtà trasformata in oneri pesanti per le famiglie, in vere e proprie tasse aggiuntive, che devono essere pagate sia per attività curricolari sia per attività extracurricolari. Riguardo a quest'ultimo aspetto, ho più volte denunciato in Commissione l'assoluta mancanza di controllo e di direttive verso i dirigenti scolastici, non ho mai ricevuto risposte. Debbo credere che il Governo, non solo non si interessi alla cosa ma, conoscendola bene, lascia che nelle scuole vengano spesi centinaia di milioni di euro, raccolti presso le famiglie, per attività scolastiche sportive, per ameni corsi di yoga, di lingua straniera, di musica, per gite, soggiorni, settimane bianche, acquisto di materiali di ogni genere, assicurazioni, perfino imposte non dovute per l'iscrizione al primo o al secondo anno delle superiori. Il tutto avviene senza contratti, senza procedure di gara per la scelta del contraente, senza il pagamento delle relative imposte, in barba alla tanto decantata lotta all'evasione. Voglio vedere se qualcosa cambierà in merito. Certamente, questo decreto‑legge è stata un'occasione mancata, perché avrebbe potuto fissare alcuni semplici principi in merito, così da orientare in modo più legale il comportamento degli istituti scolastici. *(Applausi

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, varare un decreto‑legge per l'urgenza di un regolare e ordinato avvio dell'anno scolastico il giorno stesso in cui l'anno scolastico inizia credo sia già questa una dimostrazione di una cattiva politica scolastica. Comunque, questo decreto-legge non ha impedito il prodursi di quei gravi inconvenienti che, peraltro, già in misura minore si erano verificati lo scorso anno e che quest'anno hanno caratterizzato le scuole di quasi tutte le principali città italiane (penso in particolare a Roma), con balletti di cattedre, cattedre scoperte senza docenti; veramente un disastro rispetto a qualche anno fa quando con il ministro Moratti l'anno scolastico iniziava regolarmente pressoché in tutta Italia. Devo dire che questo decreto-legge, come tutte le iniziative del ministro Fioroni, denuncia una totale assenza di strategia: siamo di fronte a una politica scolastica che risponde a delle istanze mediatiche, che interviene sulla base di stimoli del giorno per giorno, ma che è assolutamente priva di un riferimento, di valori, di una visione della società e di una concezione della scuola.

le riforme Moratti. È molto singolare come questa maggioranza, che aveva vinto le elezioni promettendo di cambiare *in toto* la riforma Moratti, ne replichi in sostanza alcuni provvedimenti, magari fingendo di abrogarli per ripresentarli come propri e quando se ne discosta certamente li peggiora.

vale ancora gli esami di riparazione: abbiamo già sostenuto che si tratta in realtà di un diverso modo di scontare i debiti scolastici che per la prima volta venne affrontato e risolto, a mio avviso in modo più equilibrato e più serio rispetto alla previsione previsione che Fioroni ha annunciato nei giorni scorsi in conferenza stampa, perché venne già introdotto dal ministro Moratti nella famosa legge n. 53 del 2003.

un autorevole giornale abbia dichiarato: peccato che il centro-destra non abbia riportato la grammatica, cioè uno studio serio della lingua italiana nelle nostre scuole; avrebbe dovuto dire qualcosa di destra. Questi stessi giornali il 9 novembre 2002 dicevano che grazie alle pressioni di Alleanza Nazionale rientrava nelle indicazioni nazionali, cioè nei programmi, uno studio più serio della grammatica, della sintassi e dell'analisi logica. È dunque evidente la carenza d'informazione e la totale totale disinformazione che attua questo Ministro. Scompare il voto di condotta; se vogliamo una scuola seria credo che un voto di condotta, nonché la possibilità di essere promossi sulla base della frequenza obbligatoria di una certa percentuale di lezioni siano

ritengo sia stato un errore, per esempio, avere riammesso la possibilità che dall'istruzione professionale si possa accedere direttamente all'università, perché corriamo il rischio di avere dei cuochi che non sapranno fare il loro mestiere o degli studenti universitari senza adeguate basi culturali.

dunque vi era anche da recuperare l'inflazione). E quei famosi 250 milioni, già stanziati dal precedente Governo di centro-destra, destinati agli incentivi, ora, dopo un anno e mezzo, vengono finalmente utilizzati per pagare il TFR. Allora, dove sta la svolta, anche in questo? Ma veniamo al provvedimento,

scuole, le classi a 40 ore erano persino aumentate con il ministro Moratti: e allora, se, per il tempo pieno, la differenza della riforma Fioroni rispetto all'andamento della scuola con il ministro Moratti consiste nella necessità delle compresenze, ci troviamo di fronte ad un'autentica presa in giro. Per quale motivo? Perché l'articolo 1 prevede che avvenga la reintroduzione del tempo pieno ad invarianza di organico, non solo, ma senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dunque, se le classi a 40 ore già esistevano prima, addirittura erano state aumentate dal ministro Moratti, e il tempo pieno significa aumento degli insegnanti nelle classi, tutto questo non sarà possibile per il vostro provvedimento. Poi ancora, sulla maturità: anche qui, vi è la presa d'atto di un clamoroso errore del ministro Fioroni. Occorre stanziare altri 45 milioni di euro, sottratti ai bilanci delle scuole: vi ricordate quando è stato dalla senatrice Acciarini che i genitori erano costretti a portare da casa persino i gessetti e le matite, perché erano stati tagliati i bilanci delle scuole? Ora, i genitori cosa dovranno fare, addirittura portare da casa i banchi, visto che continuate con questa politica di tagli ai bilanci delle scuole per finanziare una maturità che non ha certamente prodotto quei significativi risultati che in qualche modo avevate promesso? L'aumento di bocciature e una maggiore serietà della nuova maturità sono dati dalla reintroduzione degli scrutini di ammissione, già previsti nel decreto Moratti (anzi, tolti da tolti da Berlinguer, erano stati reintrodotti dal ministro Moratti): semmai, avete indebolito la serietà di questa verifica finale, perché abbiamo visto...

Dicevo che è successo che, grazie ai commissari esterni, sono aumentate del 25 per cento le rinunce e abbiamo trovato insegnanti precari a comporre le commissioni di maturità. Dunque, c'è stato un indebolimento, quanto meno sotto il profilo dell'esperienza. Poi, ancora, c'è il discorso delle valutazioni. La valutazione delle scuole, uno dei pilastri della progettualità della passata maggioranza di centro-destra: l'avete sospesa per un anno e mezzo, e noi a sostenere che era uno strumento decisivo per il miglioramento della qualità del nostro sistema scolastico;

le sanzioni disciplinari, misura senz'altro auspicabile: in assenza di un codice deontologico che fissi i doveri dei docenti credo però che rischi di risultare una misura velleitaria. Fra l'altro, avete dimenticato (e la Commissione affari costituzionali della Camera lo ha stigmatizzato) di prevedere il principio del contraddittorio. venga bocciato; la sua politica universitaria credo che venga bocciata da questo decreto-legge. Aveva promesso stanziamenti importanti per

i lavori e gli articoli di ogni singolo ricercatore italiano: ciò comporterà il fallimento della riforma della valutazione, perché impedirà all'Agenzia di valutazione di svolgere il suo compito. Caro ministro Fioroni, credo che che qui ci troviamo di fronte alla necessità di una chiara svolta culturale. Quando noi riteniamo, per esempio, che il principio di autorità debba ritornare nelle scuole e dunque, per esempio, che debbano essere tutelati gli insegnanti, prevedendo come procedibile d'ufficio qualsiasi minaccia o qualsiasi offesa alla loro dignità, lanciamo un messaggio culturale preciso; quando chiediamo che lo stipendio venga sempre più commisurato al merito, diciamo un "no" ad una scuola egualitaria, quella che voi, a partire dal '68, avete costruito. Caro ministro Fioroni, mi rendo conto che per lei è un esercizio molto difficile di politica legislativa e scolastica governare con una maggioranza così composita e disarticolata; noi, tuttavia, non ci fermeremo qua nel denunciare una politica del tutto inadeguata e del tutto falsa nelle premesse e nelle promesse.

questo decreto contiene di tutto, è un provvedimento *omnibus* che riguarda complessivamente il sistema scolastico, ma che ha la presunzione di affrontare tanti temi senza risolvere alcuno dei problemi di questo segmento fondamentale per la nostra scuola. Rilevo con profondo rammarico che, dal punto di vista della tecnica legislativa, dell'utilizzo dello strumento legislativo per risolvere problemi siamo davvero molto in basso. Utilizzando

pochissimi minuti pure in assenza di un programma organico. Poco fa il collega Amato sosteneva che il Ministro, ad inizio legislatura, affermava che avrebbe utilizzato il cacciavite: il nostro Ministro usa solo il microfono il nostro Ministro usa solo il microfono e gli effetti annuncio, dopodiché il Parlamento deve andargli appresso con i decreti di urgenza. Mi appello ai colleghi della maggioranza: fino a quando pensate che potremo parlare di scuola soltanto nel primo e nel secondo Bersani o con questo o quell'altro decreto di urgenza? Quando questo Parlamento potrà essere investito di una discussione complessiva e corposa rispetto a questo che è un settore strategico per il nostro Paese? Amici della maggioranza (mi riferisco soprattutto agli amici della ex Margherita), come è possibile che viviate la vostra vita parlamentare con un sottotitolo costante: «Vorremmo, ma non possiamo»? Voi vorreste una scuola aperta e che forma i giovani, ma non potete e quindi votate provvedimenti che vanno addirittura contro gli interessi dei diversamente abili; quei diversamente abili che si vedono negati gli insegnanti di sostegno, sostegno, quei deboli della società che andrebbero aiutati proprio lì nella scuola (perché a casa, nelle altre strutture, vengono aiutati grazie agli interventi degli enti locali): quando devono socializzare,

reintroduciamo il tempo pieno ma ad invarianza di spesa. Che vuol dire «ad invarianza di spesa»? Quando si crede nelle proprie idee, su di esse si investe; quando si crede in una strada, questa va percorsa fino in fondo. Cosa vuol dire non dare soldi alla scuola e invece volere il tempo pieno, quindi il doppio il doppio degli insegnanti e una serie di strutture che serve a rendere il tempo pieno davvero formativo, altrimenti è solo propaganda, altrimenti è solo fumo negli occhi? Non è certo di questo che abbiamo bisogno. Sarebbe davvero necessario riuscire a stemperare

che andate avanti per *slogan*? Come si fa ad avere un Governo con lo *stop and go*: un anno si fa una riforma, l'anno successivo lo stesso Governo ne propone l'abrogazione - come sottolineava il senatore Valditara - per quanto riguarda i ricercatori universitari? Come si fa a discutere con voi, che avete soltanto l'esigenza di far sopravvivere un Governo moribondo a colpi di fiducia e facendo finta di non sentire? Pur di andare avanti volete discutere in un sol colpo

Ancora una volta gli alunni sono il punto più marginale del nostro sistema scuola e il decreto di oggi lo dimostra - se ce ne fosse bisogno - nuovamente. Questa è la vostra cultura di Governo, queste sono le vostre inadeguate risposte al mondo dei giovani e della scuola.

per essere entrati puntualmente nel merito, richiamando anche molti altri problemi oggetto di discussione in altre sedi e nel Paese, segno evidente che c'è un bisogno di discutere in Parlamento - come affermava il collega Marconi - dell'universo scuola. Mi pare che in 7a Commissione il il dialogo sia già aperto e vi sia quindi la possibilità di contribuire con libertà al miglioramento delle premesse, delle condizioni per le decisioni che sono necessarie per irrobustire e dare forza al sistema di istruzione del Paese. Sul tema del tempo pieno, tempo pieno, sono stati richiamati anche altri interventi in un certo senso connessi. Al collega Amato vorrei dire che qui non si introducono gli esami di riparazione, che attengono ad un altro discorso. Tuttavia voglio sottolineare che anche la scelta per il tempo pieno è la premessa per mettere le basi perché non vi sia bisogno di quella procedura di debiti e crediti che non è soddisfacente e che attende di essere cambiata.

Sui temi importanti delle procedure, delle sanzioni disciplinari, dell'incompatibilità ambientale e degli interventi mirati, in sostanza in merito ai punti di massima gravità su cui l'ordinamento attuale non consente di intervenire adeguatamente,

alla revisione dello stato giuridico e, soprattutto, come evidenziato dalla collega Pellegatta, al riordino degli organi collegiali dove si colloca l'equilibrio tra i soggetti operanti nella scuola. consapevolezza che la libertà di insegnamento e lo stesso concetto di incompatibilità ambientale sono soggetti ai valori fondamentali della Costituzione e al ruolo della scuola, anche in relazione ai condizionamenti ambientali. Infine, a proposito

valutare l'attività dei soggetti, dei docenti tutti e dei ricercatori; così come è compito dell'ANVUR, in nome del Paese, valutare i risultati dell'attività complessiva delle università e degli enti di ricerca. In conclusione,

che mi consente di essere molto sintetica giacché esprimo una piena condivisione delle valutazioni da lei apportate, anche in risposta a numerosi interventi che i senatori hanno svolto in quest'Aula. quest'Aula. Ringrazio anche i componenti, tutti, della 7a Commissione per il lavorosignificativo che hanno svolto, sia pure in tempi molto ristretti, coerentemente con l'urgenza e l'essenzialità delle norme contenute nel decreto-legge che stiamo discutendo; norme tutte volte a consentire l'avvio dell'anno scolastico. E, come è noto al senatore Valditara, queste norme, trattandosi di un decreto-legge, sono già in vigore del momento primo della loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri e pertanto hanno già esplicato i loro effetti, che ritengo importanti, utili e positivi, per il funzionamento della scuola. La normativa al nostro esame, infatti, non intende affrontare

contenute in un disegno di legge, che è già stato approvato alla Camera e che reca «Norme urgenti in materia di istruzione», sul quale il Senato sarà chiamato ad una valutazione e ad una discussione approfondite. Quindi, le dovremo vedere in quel complesso. norme utili: quella sul tempo pieno; quella sugli esami di Stato, sia di terza media sia di carattere superiore; quella sulle sezioni primavera; quella sulla valutazione dei ragazzi; quelle sul personale docente, in particolare per rendere più efficace, rapido e rispondente alle esigenze tutto il tema delle sanzioni, pur in una attenta e accurata garanzia dei princìpi costituzionali e, in particolare, della libertà di insegnamento dei docenti. Vi è un ragionamento sul pagamento delle supplenze per maternità, che tanto ha tormentato le scuole in questo anno scolastico e che rende possibile ed efficace la modalità nuova di funzionamento delle scuole per valorizzare la loro autonomia, modalità attraverso i due grandi capitoli (che noi abbiamo chiamato capitoloni), di "budgettizzare" il funzionamento rendendo maggiormente responsabile la scuola stessa anche rispetto alla gestione finanziaria. Da ultimo, per quel che riguarda l'articolo 3, 3, comma 1-*bis*, il Governo si dichiara disponibile a rivedere quanto prima tale disposizione in un quadro normativo maggiormente organico.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione che sull'articolo 2, comma 5, penultimo periodo, sul quale il parere è di semplice contrarietà. In ordine all'articolo 1, comma 4-*ter*, il parere non ostativo è reso nel presupposto che la neutralità finanziaria sia garantita dalla determinazione in misura forfettaria dei compensi dovuti ai commissari per il complessivo espletamento degli esami di Stato, indipendentemente dal numero di prove eseguite. In ordine agli emendamenti, esprime parere non ostativo, ad eccezione che sulle proposte 1.105, 1.110, 1.111, 2.111 e 2.112, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 2.114

Deve concludere, senatore

Ne do lettura: «Impegna il Governo a tenere conto, ai fini della determinazione dell'organico relativo al tempo pieno, del numero complessivo di classi a tempo pieno attivate nell'anno scolastico di riferimento, anche per evitare il riprodursi di situazioni di incertezza e di disagio».

O questo ordine del giorno significa qualcosa - e allora è il preannuncio di un emendamento del Governo - o non significa nulla. Vorrei fosse chiaro questo problema. PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, qui ci siamo espressi e ci stiamo esprimendo impegnando il Governo, seriamente, ad essere conseguente alla alla determinazione che viene presa dal Senato, con il parere favorevole del Governo medesimo. Suppongo che il Governo sarà conseguente a questo impegno che assume davanti all'Aula del Senato.

italiani al Parlamento europeo, quindi un tema molto rilevante. Ricordo agli onorevoli colleghi che, come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ciascun Gruppo potrà intervenire per cinque minuti

Signor Presidente, la questione all'ordine del giorno è nota. Mentre oggi il numero dei seggi del Parlamento europeo attribuito a ciascun Paese è fissato dai Trattati, il Trattato costituzionale, con una norma ripresa dal Trattato che dovrebbe essere approvato a Lisbona nei prossimi giorni, rinvia il riparto alla decisione del Consiglio europeo adottata all'unanimità, sulla base di una proposta del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha elaborato nei giorni scorsi la proposta. La base per distribuire i seggi, invece di considerare i cittadini di ciascun Paese, come espressamente previsto dal Trattato, è fondata sui dati EUROSTAT relativi alla popolazione residente, includendo quindi anche gli immigrati residenti non cittadini. Noi contestiamo radicalmente questa scelta, e lo abbiamo detto espressamente ai relatori del Parlamento europeo convocati a Roma in un'audizione. Le risposte ricevute non ci hanno convinto. I relatori hanno affermato che non esistendo una nozione comune di cittadinanza l'unico criterio comune utilizzabile è quello della popolazione. Ma qui viene la questione politica che ci interessa. Perché il Parlamento europeo ha deciso con tanta rapidità? Perché la questione deve essere risolta al prossimo Consiglio europeo? Non vi è legame tra l'accordo sul nuovo Trattato e tale questione, che già oggi viene regolata in via transitoria dal Trattato sull'adesione di Bulgaria e Romania che attribuisce tra l'altro all'Italia, al Regno Unito e alla Francia lo stesso numero di seggi. L'urgenza sta in una scelta operata nel Consiglio europeo di giugno. Il Consiglio, nel dare un mandato vincolante alla Conferenza intergovernativa, ha anche espressamente richiesto al Parlamento europeo di elaborare una proposta entro ottobre. Chi si lamenta oggi dell'accelerazione impressa dal Parlamento europeo dovrebbe ricordarsi di questo passaggio, delle conclusioni del Consiglio. Al Ministro degli affari esteri bisogna ricordare che eravamo consapevoli di quella scelta, che ha inevitabilmente congiunto da un punto di vista politico due materie che giustamente devono essere trattate

A chi chiedeva una posizione dura e ambiziosa sul negoziato costituzionale disse: «Non mettiamoci nei panni dell'Italia europeista, sola contro tutti, perché questo è il modo peggiore di affrontare il negoziato». Ed ora, signor Sottosegretario, come riportano i giornali, ci troviamo soli contro tutti, in una battaglia giusta in cui noi appoggeremo il Governo nell'interesse nazionale, ma che, nell'interesse nazionale, non doveva essere legata allora alla conclusione del negoziato costituzionale. È stato quello un errore, forse una grave leggerezza che oggi paghiamo. Come una leggerezza è stata, allorché fu divulgata la proposta di Lamassoure, l'aver dichiarato, come fece il ministro D'Alema (traggo la citazione dalla stampa): «Non ci si può opporre alla demografia», avallando, di fatto, i presupposti su cui la relazione Lamassoure è fondata. Ma questo è il passato, di cui ovviamente in quest'Aula avremmo voluto chiedere conto al Ministro, che però oggi non è oggetto dell'atto di indirizzo che insieme agli altri colleghi abbiamo presentato. Noi ora vogliamo dare un messaggio chiaro di unità nazionale, su una questione che mette in dubbio un elemento essenziale del nuovo Trattato. Abbiamo voluto scrivere nel Trattato costituzionale che abbiamo ratificato che il Parlamento europeo, come il nostro Parlamento nazionale, rappresenta i cittadini. Non ci si può dunque sottrarre a questo imperativo nella distribuzione dei seggi tra i vari Paesi. Comprendiamo le difficoltà che ci sono state esposte dal relatore del Parlamento europeo, ma lo stesso Parlamento europeo ha riconosciuto, anche su nostra insistenza, che solo un riparto sulla cittadinanza sarebbe veramente rispettoso dei Trattati. La stessa soluzione che il Parlamento europeo propone è presentata come provvisoria. Se dunque si deve adottare una soluzione provvisoria lo si faccia, non seguendo l'inaccettabile criterio proposto dal Parlamento europeo, ma piuttosto iscrivendo nel nuovo Trattato, come aveva fatto saggiamente il Trattato costituzionale, nel paragrafo secondo dell'articolo 1 del protocollo sulle disposizioni transitorie, una tabella di riparto dei seggi che segua i criteri tradizionali senza alterare gli equilibri tra i Paesi stabiliti dai Trattati vigenti. Questa sarebbe una vera soluzione transitoria. È anzi la soluzione transitoria che il Parlamento italiano, in occasione della ratifica del Trattato firmato a Roma nel 2004, approvò con un voto sostanzialmente unanime. Lo dobbiamo spiegare ai nostri *partner* europei. La nostra non è una battaglia per avere uno o due seggi in più, ma è una battaglia di principio. È la battaglia di un grande Paese, orgoglioso della sua storia europeistica, che crede a un'Europa democratica e che vuole un Parlamento che rappresenti i cittadini.

dovrebbe varare il progetto di Trattato di riforma dell'Unione. Salvo novità, verrà affrontata la questione relativa al ridimensionamento numerico del Parlamento europeo. Il ridimensionamento numerico è opportuno. Il progressivo allargamento dell'Unione mette in crisi le regole e anche la composizione dei suoi organi, che furono concepiti per un'Unione Europea più ristretta. Il Parlamento ha approvato la scorsa settimana una proposta di revisione della sua composizione numerica, basata sul principio della proporzionalità degressiva

Questo criterio di ripartizione è inaccettabile. Il Trattato infatti stabilisce che «Il Parlamento europeo è composto da rappresentanti dei cittadini dell'Unione». Non c'è alcun riferimento alla popolazione residente, nel progetto di Trattato che a suo tempo ratificammo in queste Aule e nel progetto di revisione che sarà esaminato nel Consiglio europeo straordinario di domani.

In origine, ricordiamo, era prevista una parità di rappresentanza tra Italia, Francia e Germania; poi si aggiunse la Gran Bretagna e successivamente se ne distaccò la Germania, comprensibilmente, nel momento dell'unificazione. Quindi, quel criterio di parità della rappresentanza oggi investe Italia, Francia e Gran Bretagna.

la quale non sarebbe stato alterato il principio della parità della rappresentanza tra i grandi Paesi, di cui stiamo discutendo. La soluzione oggi possibile ci sembra ripercorra la stessa strada,

che si applichi al prossimo Parlamento europeo e renda possibile una più ponderata revisione della ripartizione dei seggi nel Parlamento europeo, in base ad un

una nuova finestra"). Colleghi, abbiamo ascoltato l'illustrazione delle due mozioni, largamente convergenti nelle motivazioni e nel dispositivo, che impegnano il nostro Governo ad esercitare una forte azione, in vista della riunione del Consiglio europeo che si terrà domani.

di questo dibattito per arrivare preparati domani all'appuntamento europeo, ma vorremmo che questo atteggiamento duro e intransigente fronte dei tanti problemi che riguardano la nostra Nazione in sede comunitaria. Chi si occupa di politica estera e di politica comunitaria sa che l'Italia

Nel momento in cui si può cominciare ad intervenire a cascata dall'alto sulla riduzione dei seggi del Parlamento europeo, si ha una sollevazione di scudi e non si vuole prendere atto che, invece, un ridimensionamento può anche essere la scintilla

Consiglio europeo del prossimo 18 e 19 ottobre rappresenta una tappa fondamentale del processo di riforma istituzionale dell'Unione dopo il rallentamento causato dall'esito negativo dei *referendum* francese e olandese. L'Italia sostiene gli sforzi della Presidenza portoghese affinché si raggiunga un'intesa sul progetto di trattato di riforma. Questa tempistica ci consentirebbe di tenere la cerimonia di firma del nuovo Trattato in occasione del Consiglio europeo di dicembre e ci lascerebbe un lasso di tempo sufficiente per la ratifica e l'entrata in vigore, prima delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009. Al tempo stesso, il Governo italiano è nettamente contrario alla risoluzione predisposta dai relatori Lamassoure e Severin su una possibile nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo. Non vi è alcuna contraddizione fra queste posizioni: la risoluzione Lamassoure e Severin è, infatti, essa stessa in netto contrasto con le previsioni del Trattato di riforma. Riprendendo una delle principali conquiste della Costituzione, il Trattato di riforma stabilisce, infatti, in maniera inequivocabile, che il Parlamento europeo rappresenta i cittadini dell'Unione e non i popoli dell'Unione, come avviene nei vecchi Trattati. La risoluzione Lamassoure‑Severin propone, invece, di stabilire la ripartizione dei seggi al Parlamento europeo basandosi sul criterio della popolazione residente in ciascuno Stato membro. Essa non riflette, quindi, i cambiamenti che interverranno a livello di Trattati e ne contraddice, anzi, lo spirito. Ciò premesso, l'adozione di una decisione sulla futura composizione del Parlamento in questa fase non corrisponderebbe ad una necessità giuridica, bensì ad una scelta politica, quella di dare un'applicazione anticipata all'articolo 9A. Per tali motivi, in occasione del Consiglio affari generali e relazioni esterne del 15 e 16 ottobre scorso, l'Italia ha manifestato la propria ferma opposizione ad una decisione che si basi sui meccanismi di ripartizione dei seggi del Parlamento europeo previsti nella risoluzione Lamassoure-Severin. L'Italia non desidera, tuttavia, in alcun modo porre ostacoli al buon esito della Conferenza intergovernativa e ha pertanto proposto di rinviare la decisione sulla composizione del Parlamento europeo ad un momento successivo all'adozione del Trattato di riforma. Il Governo italiano resta comunque disponibile a considerare eventuali soluzioni di compromesso che dovessero essere avanzate in occasione del vertice di domani, a condizione lo sottolineo - che esse non pregiudichino l'applicazione dell'articolo 9A, con particolare riferimento al concetto di rappresentanza dei cittadini, e non alterino, nella presente condizione, gli equilibri dei tre grandi (Italia, Francia e Gran Bretagna).

non vero nelle sue affermazioni. Non stiamo discutendo sulla riduzione dei parlamentari europei, che comunque vi sarà. Il problema è la redistribuzione, che deve avvenire, di tale riduzione: quindi, il discorso non è sul numero dei parlamentari europei, ma sul modo in cui deve avvenire questa riduzione e su chi deve ricadere. Per tutte queste ragioni, ribadisco l'opinione ed il parere favorevole del Governo sulle mozioni e il parere contrario sull'ordine del giorno*.

sul piano tecnico e giuridico. Forse, però, non è errato andare a cercare anche qualche giustificazione politica sul perché l'Italia oggi si trovi a dover recuperare un *deficit* nei confronti di altri Paesi, come ad esempio il Regno Unito e la Francia, con cui ha diviso, in tutti questi anni, una parità nel numero di rappresentanti al Parlamento europeo. Va detto che il calo è fisiologico, inevitabile - come ha sottolineato il Sottosegretario - perché sia il Parlamento europeo, sia la Carta costituzionale (oggi in parte degradata al rango di semplice revisione di Trattato) hanno deciso di porre a 750 il tetto massimo dei rappresentanti al Parlamento europeo.

15 rappresentanti in meno. Ciò - lo ribadisco - era fisiologico e il nostro pianto è da concentrare soltanto sui deputati europei che vengono a mancare (cioè sulla differenza di due). Quindi, 72 rispetto ai 74 che riteniamo di dover raggiungere. È stato anche chiarito che c'è una

La diatriba è tutta qui. Vincere questo braccio di ferro significa automaticamente riottenere due parlamentari in più, riconquistare la parità con Francia e Gran Bretagna, e, in caso di annessione della Turchia, riuscire anche a contenere la rappresentanza turca, che sarebbe uguale a quella italiana. Per un Paese fondatore chiaramente non vi è soltanto un motivo politico, ma c'è anche una questione di prestigio da riequilibrare. Come mai siamo finiti in questa brutta situazione? Le cronache di Palazzo, quelle un po' maliziose, riportano che il giorno in cui, nel Consiglio di primavera a Bruxelles, si decise su questa distribuzione, il nostro presidente del Consiglio Prodi si era assentato dall'Aula. Era in un corridoio preso da una interminabile telefonata con l'Italia ed impegnato soprattutto a dirimere una questione di politica interna (diciamo pure di carattere governativo) e ciò lo aveva distratto dal tema che si stava discutendo all'interno del Consiglio. Non è nemmeno esclusa l'ipotesi di una imboscata, di un trabocchetto: qualcuno, ad arte, visto che mancava il Presidente del Consiglio italiano, ha posto la questione all'ordine del giorno e ha fatto rapidamente approvare quella decisione. decisione. Cosa ci resta da fare, ora? Si può recuperare, signor Presidente, chiaramente non minacciando di non firmare il Trattato costituzionale (sarebbe deprimente per un Paese fondatore come l'Italia) e nemmeno andando a cercare (come pare stia facendo il Governo)

Presidente, come era stato illustrato prima dal collega Morselli, voteremo contro le mozioni in cui si propone di opporsi alla proposta europea di ridurre i parlamentari

che non farà che aumentare il distacco fra il Paese e la politica, perché sarà notata da centinaia di migliaia di agricoltori: ci si impegna in Parlamento contro la Comunità europea che vuole ridurre i parlamentari e non ci si impegna in Parlamento per quanto riguarda alcuni aspetti clamorosi della politica agricola. Inoltre, il Parlamento è impegnato allo stremo per non farsi ridurre i parlamentari europei e poco o nulla è impegnato

cioè il lavoro avventizio, che sta impedendo la raccolta, ad esempio, delle olive in Puglia: su questo problema si discute poco o nulla e invece ci si impegna per non ridurre i parlamentari europei. Voteremo quindi convintamente contro

deve sapere ciò che avviene, come ci comportiamo in Parlamento su questi problemi secondari e come trascuriamo invece i problemi principali della nostra

il Gruppo Per le Autonomie condivide le mozioni presentate, sia nei contenuti che nelle motivazioni, e si complimenta con i proponenti per la sostanziale condivisione e convergenza da parte di senatori della maggioranza e dell'opposizione, sostenuti anche da senatori illustri della Repubblica. Un voto a favore affinché il Governo abbia una ampio mandato da questa Assemblea per rivendicare un diritto sancito dai Trattati europei. europei. Sottolineo la valenza politica della questione, che porrebbe l'Italia in una condizione di rappresentanza inferiore a Paesi che con essa sono stati fondatori dell'Unione Europea ed hanno contribuito insieme in modo determinante alla sua crescita e al suo sviluppo. Oggi l'Europa si prepara ad approvare una importante riforma istituzionale, la firma del Trattato; un passo rilevante, anche se non soddisfa appieno le nostre aspettative di europeisti convinti. Tali sfide possono essere vinte solo se l'Europa si avvicina di più ai cittadini, favorendo tutti gli strumenti di partecipazione e di condivisione. C'è bisogno di maggiore democrazia e i Parlamenti sono le sedi rappresentative più immediate, più dirette, meglio percepite dai cittadini. Riteniamo pertanto fondamentale una equa ripartizione della rappresentanza dei vari Paesi al Parlamento europeo. Questo importante dibattito mi porta a fare alcune considerazioni sulla necessità che l'Italia, che giustamente rivendica i suoi diritti, garantisca con la sua legge elettorale una rappresentanza dei cittadini che tenga in debita considerazione le proprie articolazioni regionali e garantisca in Europa la rappresentanza delle minoranze costituzionalmente riconosciute al suo interno. In questo senso, a firma dei senatori della Gruppo Per le autonomie, è stato presentato un disegno di legge che introduce modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri della Parlamento europeo spettanti all'Italia, quale la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione autonoma Valle d'Aosta formano una circoscrizione elettorale e ad ognuna è assegnato un rappresentante.

per senso di responsabilità sosterremo lo sforzo del Governo in questa direzione, anche se siamo assai in disaccordo sul concetto di cittadinanza espresso da entrambe le mozioni.

e assumere lo *ius soli*. È la determinazione geografica e temporale che rende possibili il patto di convivenza, le relazioni, la scommessa comune. È l'abitare un luogo, il viverci, che dà valore a diritti e doveri e legittima, quindi, il concetto di appartenenza e di cittadinanza.

Dovremo chiederci se abbia senso o meno che gente che non abita più qui, che non paga le tasse, abbia la rappresentanza di questo territorio. Dovremmo, forse, concepire la cittadinanza come relazione tra persone che vivono, lavorano, si amano e litigano, ma che nello stesso territorio contribuiscono alla costruzione del patto sociale, alla ricchezza collettiva e alla ricchezza culturale multietnica. In sostanza, crediamo si tratti di una battaglia di retroguardia e chiediamo al Governo

sembrerà strano, ma a volte i più sofisticati piani si infrangono sulle più grandi banalità,

poltrone per ospitare eurodeputati. I trattati susseguenti hanno stabilito pertanto di non andare oltre, anche perché fisiologicamente non si poteva, e hanno comportato una revisione dell'originaria partecipazione e della numerica distribuzione dei seggi dell'Europarlamento.

Consiglio, il Parlamento è entrato con sempre più forza ed importanza ed il suo ruolo ha pesato sempre più nel processo formativo degli atti della Comunità. A questo punto, i numeri del Parlamento hanno acquisito una certa importanza.

del Trattato recita che: «Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti di cittadini dell'Unione», "cittadini" ha un significato.

facciamo votare e contare in Europa i Paesi con più alta densità di stranieri extracomunitari. Praticamente conteranno conteranno di più in Europa quei Paesi che hanno minore identità europea! È un'aberrazione per i princìpi costitutivi della nostra Comunità.

Dare la cittadinanza significa ammettere a far parte di una comunione spirituale - senatore Silvestri - che non è razziale, è razziale, ma di cultura. Un italiano può avere la pelle nera, ma deve amare Dante, il Tricolore e sentirsi partecipe della storia e della cultura italiane. Magari deve anche mangiare gli spaghetti. La cittadinanza è cosa diversa dalla residenza

della esistenza di scaglioni di Nazioni che dovrebbero avere uguale rappresentanza. Con il Trattato noi facciamo un grosso passo avanti, proprio perché rinunciamo a questo principio. In uno Stato federale - e noi speriamo in una Europa federale;

dei popoli ed è il Senato, oggi Consiglio dei ministri, e c'è una rappresentanza dei cittadini, che è il Parlamento, la quale deve essere basata sul principio «un uomo, un voto».

ma dovendo adottare un criterio provvisorio ha molto più senso adottare quello della somma di coloro che sono abilitati al voto nelle elezioni europee nei diversi Paesi. In questo momento la cittadinanza europea è definita dai diversi Paesi. La somma comune degli elettori si ottiene facendo la somma dei cittadini che hanno diritto al voto. È un criterio approssimativo? Sì, lo è, anche perché non considera il peso dei minori dei minori che hanno diritto di essere rappresentati tramite i loro genitori e nella definizione dei collegi elettorali bisognerebbe tenerne conto. Tuttavia, è un criterio meno imperfetto di quello che è stato adottato e andrebbe seguito in attesa di poter definire un criterio comune di cittadinanza e di elaborare anche strumenti statistici che diano una rappresentanza adeguata alla cittadinanza europea. Credo che dobbiamo insistere su questo fatto, su questo spiraglio apertosi all'interno della risoluzione. Credo che il Governo debba porre nettamente l'accento anche sul fatto che non esiste una connessione necessaria tra l'approvazione del Trattato e la soluzione di questo problema. Sono due questioni distinte. Ognuno capisce che esiste un legame fra le due questioni, ma non si può dire che non è possibile approvare il Trattato se non si risolve contemporaneamente anche questa questione. È possibile, infatti, andare a votare anche sulla base di criteri che applicano la riduzione dei rappresentanti e che sono stati approvati in precedenti Consigli europei. Presidente, mi consenta infine di fare un appunto al Governo. L'Europa è un meccanismo lento ma spietato. Quando approva un principio, si è poi tenuti a seguirne le conseguenze. Il Governo non ha tempestivamente visto la portata di questo problema. Ha dato l'impressione di potersi rassegnare a quella decisione. Ha inizialmente difeso la causa italiana con argomenti inadeguati, l'idea della parità che è esclusa dai criteri già contenuti nel Trattato. Solo alla fine ha capito e ha preso una posizione ferma. Questo ovviamente danneggia la nostra posizione negoziale. Noi invitiamo il Governo ad approvare il Trattato e a non approvare questo regolamento di voto.

dato al Governo in questi passaggi e quindi il dispositivo delle mozioni, ma credo che anche su questa questione alcune considerazioni che in qualche modo ci diversificano vadano fatte. fatte. La nostra contrarietà e la nostra opposizione alla proposta di nuova ripartizione dei seggi del Parlamento europeo non ha infatti come punto centrale ed esclusivo la difesa, che pure riteniamo legittima, del ruolo del nostro Paese all'interno della Comunità europea. Non nasce esclusivamente da un giudizio sulla ingiusta penalizzazione dell'Italia che ha più di altri - come tutti sappiamo - sostenuto con convinzione e coerente continuità lo sforzo di costruzione di una Europa unita e solidale, una Europa dei popoli come noi diciamo. Nemmeno le nostre argomentazioni si limitano ad interpretazioni giuridiche sulla lettera dei trattati che pure hanno una loro evidente attendibilità. Il cuore del problema crediamo sia un altro - è l'elemento centrale della nostra opposizione alla proposta votata a maggioranza l'11 ottobre scorso - e sta nel valore irrinunciabile che intendiamo attribuire al Parlamento europeo, nella convinzione che esso debba funzionare come concreto ed efficace strumento della rappresentanza; una efficacia che non può che basarsi sul rispetto, signor Presidente, dei principi basilari, a partire dalla natura soggettiva del diritto di espressione del voto e della sua capacità di contribuire al pari degli altri aventi diritto alla formazione della Assemblea elettiva. Affinché ciò si realizzi è indispensabile che vi sia una relazione diretta tra il numero dei votanti e quello dei seggi attribuiti; che vi sia una analoga platea destinata ad individuare il numero dei rappresentanti e coloro che ne hanno diritto al voto. Se si rompe tale relazione, di fatto si assegna a qualcuno il potere di decidere per altri, ai votanti la possibilità di decidere per i residenti non votanti, stabilendo così inaccettabili gerarchie nei diritti. Altra questione - tutt'altra questione non è questa purtroppo sollevata nella determinazione europea - è l'allargamento della cittadinanza e l'universalità del diritto al voto, su cui è invece necessario impegnarci ciascuno nel proprio Paese fino a che questa rimarrà esclusiva materia delle comunità nazionali. Su questi temi ci siamo espressi con chiarezza nel senso dell'allargamento dei criteri di cittadinanza, nel superamento di quell'iniquo e medievale *ius sanguinis* che definisce ancora il diritto e la possibilità di accesso alla cittadinanza. Solo i principi della democrazia, del suo allargamento e del rafforzamento dei suoi strumenti possono guidarci in questo passaggio combinando i diritti individuali - il diritto di voto - con l'esigenza di modulare la rappresentanza per garantire le minoranze politiche ed i piccoli Stati che entrano e che sono parte oramai dell'Europa. Il Consiglio straordinario di Lisbona del prossimo 18 ottobre affronterà la questione ed avrà come compito quello di trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di modificare l'impostazione uscita dalla precedente riunione e l'esigenza di non ricorrere al diritto al veto, e noi riteniamo comunque un esercizio non costruttivo e non corrispondente ad un corretto esercizio del confronto. Rinviare ogni decisione all'annunciata revisione delle modalità di piena attuazione del suffragio universale (su cui dovremo lavorare, nel senso che qui abbiamo detto), in vista poi del rinnovo del Parlamento del 2014, è, non solo un giusto obiettivo che ci sentiamo di sostenere, un obiettivo politico, ma è anche un ragionamento dotato di forte razionalità, di capacità di convinzione e che ci può mettere sul terreno di una concreta evoluzione dell'organizzazione della rappresentanza, che non può essere sottoposta allo *stress* di un continuo cambiamento, in forza del quale si fa un criterio, poi se ne fa un altro nel 2009 ancora nel 2014. È lì che noi dovremo traguardare, sia per quanto riguarda il nostro impegno nazionale di allargamento del criterio di cittadinanza, di avvicinamento dei concetti di popolo, di cittadini e di votanti, sia per quanto riguarda il complessivo approccio del Parlamento europeo e delle Istituzioni comunitarie.

dire al Governo, con grande serenità, che le due mozioni nel loro dispositivo impegnano il Governo a non dare il proprio consenso. Vorrei che fosse capito l'auspicio di una posizione forte che il Governo deve assumere domani e dopodomani a Lisbona: non si tratta, cioè, di un mandato da parte del Parlamento ad assumere un atteggiamento deciso, ma in qualche modo in quella sede conciliabile. O in quella sede si torna alla proposta dei 736 come numero totale dei membri dell'Assemblea dell'Assemblea o si ripristina la parità di peso tra Francia, Italia e Inghilterra (che è un'antica tradizione del Parlamento europeo), oppure non si dà il consenso, rimandando ad altro tempo, ovviamente, l'ipotesi di soluzione, ma dimostrando che il Governo italiano su questo argomento non è disposto ad infrangere dei princìpi che sono insiti nella vicenda parlamentare europea. Dico perché mi rendo conto della difficoltà del Governo e forse questo spiega anche le difficoltà o i contrasti tra maggioranza e opposizione. C'è sempre stata l'accusa, da parte del centro‑sinistra al centro‑destra, di non credere nell'Europa, di essere euro-scettici o di non avere nei confronti dell'Europa un atteggiamento aprioristicamente positivo. Noi diciamo - e questa ne è la conferma - che si partecipa all'Europa per costruire una grande Europa, ma che i problemi dell'interesse nazionale sono sempre all'attenzione quando si tratta in Europa. L'Europa è una grande famiglia, ma non per questo i fratelli, i cugini, i parenti sono sempre disponibili a comprendere le nostre posizioni e le nostre valutazioni. Questo rapporto con l'Europa va definito una volta per tutte con grande chiarezza: si è all'interno dell'Europa per costruire una grande Europa, nel rispetto di quelli che sono gli interessi nazionali. contrario vivremmo una vicenda che abbiamo vissuto per molto tempo - dall'acciaio all'agricoltura - in cui le ragioni degli altri, siccome sono europee, devono sempre prevalere sulle nostre. Ci sarà pure una ragione se il presidente Sarkozy ha anche deciso di non compiere il gesto che gli era stato chiesto, ossia di rinunciare ad un seggio per ripareggiare la questione. Evidentemente, nella concezione francese, il fatto che il Paese abbia 74 seggi, e che quindi appaia, anche nell'immaginario collettivo, come il Paese più importante del Parlamento europeo, dà un significato alla politica che il Presidente francese persegue. Così come gli altri hanno questi problemi, anche noi abbiamo il nostro, che è quello di essere considerati tra i tre grandi Paesi dell'Europa: Gran Bretagna, Francia e Italia. Gran Bretagna, Francia e Italia. Dico questo perché non vorrei che questo passaggio parlamentare - ringrazio la sensibilità della Presidenza, che ha voluto questo dibattito inserito il giorno prima dell'incontro di Lisbona - fosse assunto come una delle tante raccomandazioni o delle tante perorazioni che il Parlamento rivolge al Governo. Credo che il Parlamento italiano oggi, esprimendosi sostanzialmente in senso unanime, al di là di come andranno i meccanismi di voto, dice chiaramente al Governo: in Europa sì,

al Senato che anche oggi, tanto per ripetere questo triste rito, nella Regione Lazio, qualche ora fa, nel cantiere dell'ENEL di Torre Valdaliga Nord, corso la trasformazione del vecchio impianto a carbone, è avvenuto un altro incidente mortale: è morto un giovane, schiacciato da un tubo.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, egregi colleghi, credo che la vicenda sia stata esplicitata con chiarezza dai senatori intervenuti prima di me. Da parte mia voglio solo riassumere brevemente quel che penso sul piano politico essere un dato negativo per il nostro Paese. Il Consiglio europeo di giugno aveva dato mandato al Parlamento europeo di formulare una proposta sulla composizione del Parlamento stesso, entrasse in vigore a partire dal 2009. Tale proposta è stata votata dal Parlamento europeo e vede per la prima volta - questo è un dato storico - il nostro Paese rappresentato con un numero di parlamentari inferiore a quello degli altri Paesi europei omologati al nostro, cioè la Francia e la Gran Bretagna. Avremmo, quindi, un europarlamentare in meno se questa proposta fosse fatta propria dal prossimo Consiglio europeo. Il documento che abbiamo presentato sta proprio a significare la nostra contrarietà rispetto al voto del Parlamento europeo. Chiediamo quindi al Senato di sostenere questo documento che abbiamo presentato, e che a nostra volta sosterremo, per quanto riguarda il dispositivo della proposta, firmata anche dai colleghi Dini ed altri, che prevede che nel Consiglio europeo prossimo venturo il Governo italiano non acconsenta a sostenere una proposta irricevibile. Lo è perché anche sul piano giuridico - è stato ricordato - non tiene in considerazione un principio fondamentale, quello della cittadinanza, ma prevede viceversa che il numero di parlamentari venga edotto dalla residenza all'interno dei singoli Stati membri. Lo stesso Parlamento europeo ha dichiarato questa come proposta provvisoria, essendo l'unico elemento oggi sul

giusto, più corretto. L'unico parametro giusto e corretto è quello della cittadinanza. È del tutto evidente. I Parlamenti sono rappresentanza della cittadinanza e non certamente della residenza. Siamo quindi a chiedere di non sostenere questa proposta. Vogliamo con questo voto, congiunto a quello della maggioranza, dare forza al nostro Governo, perché non sia minimamente disponibile ad accettare tale penalizzazione. Credo però sia giusto da parte nostra fare anche un'osservazione di tipo politico. Questa non vuole essere una polemica, ma penso sia anche corretto fare qualche piccola osservazione. La domanda che faccio ai colleghi della maggioranza e al sottosegretario Crucianelli è la seguente: se, *mutatis mutandis*, questa proposta fosse stata fatta quando al Governo c'era l'onorevole Berlusconi, secondo voi, cosa sarebbe successo nei *mass media*, cosa avrebbe fatto l'attuale maggioranza, quali sarebbero stati gli atteggiamenti che voi avreste assunto?

avevamo distrutto l'immagine dell'Italia e che eravamo stati capaci di essere dileggiati anche a livello internazionale. Bene, questa accusa noi a voi non ci sentiamo di farla, perché abbiamo a cuore

cui tutti noi potessimo riflettere e che tutti facessimo tesoro di questa proposta, per evitare in futuro che questioni di interesse generale possano essere assunte strumentalmente per addossare la colpa

il voto favorevole del Gruppo Ulivo alle identiche conclusioni delle mozioni accettate dal Governo, ha tre precisi In primo luogo, è la difesa della certezza del diritto nell'ordinamento costituzionale europeo. Sappiamo benissimo che si tratta di un ordinamento in costante evoluzione, ma siamo anche convinti che ogni programma di progresso giuridico non può basarsi su rotture di sistema. Ogni progresso deve svilupparsi su basi precise di diritto e la stessa forza propulsiva di un ordinamento deve trovare la sua legittimazione su chiare clausole evolutive. Non c'è posto per improvvisazione ed anarchia, vizi che sono purtroppo dietro alla decisione del Parlamento europeo, che con grave disinvoltura, ha mutato il parametro di riferimento della rappresentanza parlamentare, spostandolo dal criterio di cittadinanza a quello di residenza. Certo, le regole di cittadinanza sono mutevoli da Paese a Paese e un'armonizzazione è da augurare. Ma, prima di questa armonizzazione, la regola costituzionale è che, come dicono i trattati vigenti, "la cittadinanza europea completa quella nazionale" ma "non si sostituisce" ad essa. Questa rimane l'unico riferimento possibile nel mondo del diritto per la rappresentanza politica, ed essa non ammette deroghe, neppure provvisorie. Ricordiamo che, in passato, per concedere la possibilità di voto amministrativo alcuni Stati hanno dovuto cambiare addirittura la loro Costituzione; figuriamoci se facilonerie sono accettabili quando l'elezione riguarda la rappresentanza politica europea. La seconda ragione è che la decisione del Parlamento europeo non ha né la legittimazione, né la natura per entrare a far corpo con il nuovo trattato di riforma, quello che i Governi sono in procinto di approvare. Non ha la legittimazione perché è stata presa sulla base di una norma che non è ancora entrata in vigore (il famoso articolo 9A), ma solo nell'ipotesi che essa entri in vigore. Non ha la natura del trattato con cui si vorrebbe accoppiare, con una forzatura inammissibile: perché la procedura di revisione, in ogni sua parte, secondo i trattati vigenti, deve seguire un percorso che è variabile soltanto con la stessa procedura. Siamo infatti in presenza della norma di chiusura di ogni ordinamento. Una norma fatta di regole precise: una convenzione parlamentare in cui c'entrano i Parlamenti nazionali, la Conferenza intergovernativa, il voto unanime. Sono tutti requisiti che qui non non riscontriamo. E non si tratta di un protocollo addizionale o sussidiario. La terza e ultima ragione è di natura più politica. Possiamo comprendere che una maggioranza di colleghi del Parlamento europeo (anche se ben 263 parlamentari hanno votato contro o si sono astenuti) auspichi che la rappresentanza al Parlamento europeo tenga conto del peso demografico, sociale e politico di quelli che, senza essere cittadini, convivono tuttavia nel territorio di uno Stato. Ma proprio per questo nostro pregiudizio favorevole ad un allargamento del recinto della rappresentanza politica, sappiamo benissimo che una materia come questa, in radicale mutamento rispetto a una delle ultime ridotte dello Stato nazionale, impone - come hanno detto i senatori Silvestri, Mele e Allocca - una riflessione altrettanto radicale sul modo di essere dell'Unione e degli Stati nazionali in essa. Non è certo materia

come una nostra dissociazione dall'approvazione della riforma del Trattato, che è il modesto risultato che possiamo raccogliere dopo le delusioni per lo stallo del processo costituente. vista la sua benevolenza, che questa motivazione, a mio avviso, sarebbe stato bene scriverla non soltanto nelle premesse, ma nel dispositivo della mozione. *(Applausi dei senatori Zanda

che se solo il senatore Giannini, dopo aver chiesto al prefetto e al sindaco un incontro urgente, avesse usato la cortesia istituzionale di presenziarlo personalmente, senza lasciare soli il segretario e i dirigenti di Rifondazione Comunista, saprebbe intanto che l'ordinanza emessa, e non ancora eseguita né notificata, risponde a profili di responsabilità ineludibili, per un immobile, fra l'altro, non ancora a norma. Tuttavia il problema resta. Quando esistono 700 domande di assegnazione di alloggi, di cui 200 di grave emergenza, e quando il Comune fronteggia già con fondi propri il problema del fitto per 100 di queste famiglie, non è possibile per nessuno privilegiare solo quelli che occupano gli immobili e/o solo le famiglie del Comitato organizzato dai locali dirigenti di Rifondazione C'è bisogno di risorse e in tale direzione potrebbero dare un contributo fattivo, concreto e urgente sia il Ministro per la solidarietà sociale sia l'assessore regionale calabrese per